L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

quello della garanzia per tutti di una convivenza civile, che è obiettivo primario dell'azione del Governo, come dimostrano i primi provvedimenti licenziati la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, e su un profilo di carattere più specifico, i rom, sui quali i lavori sono in corso nei termini che saranno esposti tra breve. Come ha affermato il Ministro dell'interno in occasione del 156° anniversario della Polizia di Stato, per evitare che la rabbia prevalga sulle regole della convivenza e che si ripetano episodi di violenza ingiustificabile come quelli di Napoli, è necessario intervenire con fermezza per contrastare la sfiducia nelle istituzioni e per dare risposte convincenti al senso di insicurezza dei più. Ribadisco quindi la condanna netta e senza riserve delle violenze e delle intolleranze contro i rom registrate nelle settimane scorse - e anche negli ultimi giorni in alcune località della nostra Nazione e, al tempo stesso, la volontà del Governo di agire con determinazione per rimuovere le cause che sono a monte delle manifestazioni di intolleranza. La tutela delle popolazioni rom si realizza non militarizzandone gli insediamenti per difenderli da eventuali attacchi, ma evitando che esse siano percepite, a torto o a ragione, come una minaccia per la sicurezza delle nostre città. Vanno quindi anzitutto distinti i rom che delinquono da quelli che rispettano le regole: i primi vanno perseguiti col rigore dovuto indifferentemente agli italiani e agli stranieri che si pongono contro le leggi dello Stato; gli altri devono essere aiutati a proseguire un percorso di integrazione e di inserimento sociale che non può prescindere dal rispetto delle norme. Per quanto riguarda in particolare i fatti di Napoli, l'area partenopea ospita un numero elevato di famiglie rom di etnia slava e rumena che vi si sono insediate con modi e in tempi diversi: quelli provenienti dalla ex Jugoslavia (per lo più concentrati fra Secondigliano e Scampia), presenti da oltre vent'anni, e quelli di origine rumena, insediatisi prevalentemente a partire dal 2002. Secondo i dati forniti dalla prefettura di Napoli, la presenza in provincia si aggira complessivamente sulle 5.400 unità, di cui circa 800 nei campi attrezzati dal Comune ubicati nell'area retrostante il carcere di Secondigliano e altri 120, tutti provenienti dalla città rumena di Calarasi, sistemati presso l'ex scuola Deledda. Agglomerati spontanei ed abusivi si trovano nei quartieri napoletani di Ponticelli, Scampia, Poggioreale e Pianura, dove vivono complessivamente circa 2.000 rom. Nel quartiere Ponticelli, in particolare, risultano censiti sette insediamenti spontanei, con una presenza complessiva di 600 persone rumene provenienti dalla regione moldava. In provincia, i maggiori insediamenti si trovano a Giugliano, Caivano, Torre Annunziata, Acerra, Nola, San Giorgio, Casoria, Torre del Greco e Afragola-Casalnuovo. I nomadi presenti in questi insediamenti abusivi vivono in un contesto di degrado socio-ambientale caratterizzato da differenti manifestazioni di devianza sociale. mentre i capi famiglia sono dediti prevalentemente al commercio minuto, alla raccolta di metalli e al lavoro edile, gli altri sono abitualmente impegnati nella pratica dell'accattonaggio ed in forme tipiche di criminalità diffusa, quali i furti negli appartamenti e presso gli esercizi commerciali, che incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Conseguentemente, i rapporti tra i rom e la comunità residente nel quartiere di Ponticelli a Napoli, all'origine improntati alla tolleranza, si sono progressivamente deteriorati soprattutto a causa dell'incremento degli insediamenti, che hanno inciso sul degrado urbano della zona, anche sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie, oltre che della sicurezza. Ad innescare i fatti delle scorse settimane, come tutti sanno, è stato l'episodio avvenuto il 10 maggio, quando una rom minorenne è stata arrestata con l'accusa di essersi introdotta illecitamente in un appartamento di via Principe di Napoli, nelle vicinanze del campo nomadi di via Malibran, e di avere tentato di sottrarre una bambina di sei mesi alla madre. La vicenda ha determinato la reazione di parte dei residenti della zona che, nella notte successiva, hanno lanciato bottiglie incendiarie verso il campo ubicato in via Petri, provocando la distruzione di alcune baracche. Al verificarsi di tali eventi il questore di Napoli ha disposto il potenziamento delle misure a protezione di tutti gli insediamenti dei nomadi, anche attraverso l'impiego di decine di unità del reparto mobile della Polizia di Stato. La situazione dell'ordine pubblico si è aggravata il 13 maggio quando, in coincidenza con le riprese della trasmissione RAI «La vita in diretta», centinaia di persone si sono radunate nelle vie principali del quartiere Ponticelli dando luogo a blocchi stradali, mentre un gruppo di residenti ha tentato di penetrare nel campo nomadi di via Malibran. Il tempestivo intervento degli operatori di polizia ha impedito il contatto fisico tra le parti, ma non il lancio, a distanza, di pietre all'indirizzo dei rom. Nonostante i servizi di vigilanza predisposti, approfittando dell'oscurità, dei malintenzionati sono riusciti ad appiccare il fuoco ad alcune baracche sia al campo nomadi di via Malibran, in prossimità di via Argine, sia al fabbricato in disuso - ex sede dell'istituto Tropeano - di via De Meis. Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza ed evitare che l'onda d'intolleranza si propagasse all'intera provincia, sono state attivate le forze dell'ordine per predisporre dispositivi preventivi a tutela delle persone che vivono negli accampamenti, intensificando anche l'attività informativa in modo da acquisire per tempo notizie sull'eventuale preparazione di altri attacchi e modulare conseguentemente la predisposizione dei relativi servizi. Particolare attenzione è stata rivolta a verificare la presenza di minori abbandonati e ad attivare, anche attraverso la protezione civile, misure di assistenza e ricovero in favore di alcune decine di bambini. Si è inoltre ritenuto opportuno ospitare i rom residenti nel quartiere nel campo principale di via Malibran e, successivamente, su indicazione dell'Opera nomadi, la maggioranza di essi si è allontanata dalla zona per raggiungere insediamenti ubicati fuori Comune oppure nel centro di accoglienza di via Santa Maria del Pianto, nel quartiere Poggioreale. Nella mattinata del 14 maggio altri appartenenti alla medesima etnia hanno lasciato il quartiere ove, nel primo pomeriggio, un gruppo di circa 50 persone, composto prevalentemente da donne, ha effettuato un ulteriore blocco stradale in prossimità di uno dei campi, dove gli ultimi nuclei familiari rom erano ancora in attesa degli automezzi messi a disposizione dall'amministrazione comunale per il loro trasferimento. Alcuni ricoveri del campo di via Calibra, già completamente abbandonato, sono stati parzialmente incendiati da ignoti, che sono stati messi in fuga dalle forze dell'ordine in servizio di vigilanza nella zona. Queste ultime, su segnalazione di un operatore televisivo presente sul posto, hanno poi rinvenuto, in prossimità dell'insediamento di via Malibran, due bottiglie incendiarie occultate. Tutto ciò ha indotto a collocare un presidio fisso delle forze dell'ordine in quelle strutture per evitare nuovi episodi di violenza e di intolleranza. Nell'ambito dei servizi di vigilanza disposti operatori di polizia hanno anche sorpreso e tratto in arresto due giovani, intenti a rubare un generatore di corrente all'interno di uno degli insediamenti. Infine, un nuovo episodio illecito si è verificato ieri mattina nel campo abbandonato di via Virginia Woolf, a Ponticelli, dove, intorno alle 9, un incendio appiccato da ignoti ha danneggiato baracche e masserizie. L'intervento dei vigili del fuoco e del personale del commissariato di polizia ha consentito di spegnere l'incendio, domato alle ore 11,30. Sui fatti del 13 e 14 maggio la DIGOS di Napoli ha inoltrato all'autorità giudiziaria un'informativa che riepiloga la prima attività svolta. Sulla base degli elementi investigativi finora raccolti dagli inquirenti non emergono al momento ma vorrei sottolineare al momento - elementi che comprovino ingerenze della criminalità camorristica nell'organizzazione o nella gestione delle aggressioni, né collegamenti con gruppi politicizzati o del mondo antagonista; e ciò benché, in un'analisi di scenario, non si possa escludere che la criminalità locale, strumentalizzando l'insofferenza che serpeggia fra la popolazione, possa cavalcare le proteste xenofobe per affermare la sua presenza sul territorio. La questione è all'attenzione delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia che, per garantire una più efficace azione di prevenzione generale, dispongono e rivedono periodicamente, in sede di coordinamento tecnico, le strategie per garantire, da un lato, un più capillare controllo del territorio, con priorità dei servizi di sorveglianza sugli obiettivi più esposti a rischio, dall'altro, l'intensificazione dell'attività di informazione preventiva per la rilevazione costante di ogni situazione di pericolo. L'attività di prevenzione mira ad incidere con determinazione sulla complessiva attività criminale nella Regione, che nel corso del 2007 ha registrato oltre 230.000 delitti, con più di 76.000 persone denunciate, delle quali 18.608 in stato di arresto. Di tali delitti, 533 sono riconducibili a persone di nazionalità ex jugoslava e 951 a persone di nazionalità rumena. Infine, nell'ambito dei provvedimenti in materia di sicurezza approvati dal Consiglio dei ministri a Napoli nella seduta del 21 maggio, accogliendo la richiesta di urgente adozione di misure eccezionali formulata dal Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato fino al 31 maggio 2009 lo stato di emergenza in relazione all'insediamento di comunità nomadi nel territorio delle Regioni Campania, Lombardia e Lazio. Attraverso l'emanazione di ordinanze di protezione civile e con il diretto coinvolgimento dei prefetti di Roma, Milano e Napoli sarà possibile far fronte con rapidità alle situazioni più critiche determinate in quelle aree. La messa a punto degli aspetti operativi del provvedimento è stata oggetto anche di un incontro che si è svolto il 22 maggio al Viminale alla presenza, tra gli altri, del Ministro dell'interno, del Sottosegretario con delega all'emergenza rifiuti, del presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, dei sindaci di Roma e Milano, dell'assessore delegato dal sindaco ai servizi sociali del Comune di Napoli, oltre al capo della polizia, ai prefetti di Roma, Milano e Napoli

il nostro. Per non dilungarmi, in assenza di tempo, cito la presa di posizione dei rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio, che pongono in evidenza il vero punto essenziale della complessa problematica dei rom e dei gruppi assimilabili.

Sono preoccupato del fatto che si dichiari uno stato di emergenza per i rom e categorie assimilabili di cittadini stranieri, se questo stato di emergenza non vedrà il suo fulcro in un programma di inserimento e di reale predisposizione di quelle condizioni indispensabili affinché i rom e altri cittadini stranieri, che sono persone come noi,

le baraccopoli di rom e altre comunità creano disagi e problemi, a loro stessi ma anche ai cittadini che subiscono determinate conseguenze, ma limitare l'intervento al momento repressivo significa reiterare la nostra incapacità, la nostra disfatta nei confronti di queste persone e dell'intero problema. Non ho difficoltà a ricordare anche le responsabilità del Governo precedente. Ci viene ricordato giustamente che in Italia non abbiamo utilizzato i fondi dell'Unione europea per questo tipo di programmi. Allora, in questo clima - che apprezzo - di predisposizione alla collaborazione

accingo a rispondere riguardano alcune importanti infrastrutture ricadenti nel territorio bolognese, che rivestono un'importanza strategica per lo sviluppo regionale e che sono fortemente sentite e volute da tutte le realtà economiche e amministrative dell'area interessata. Desidero qui assicurare, naturalmente, che il Governo ha costantemente presenti gli interessi di tutte le Regioni italiane, dalle Alpi alla Sicilia, tanto più se trattasi di aree economicamente e produttivamente rilevanti quali appunto l'Emilia Romagna. È bene ricordare, e l'occasione che si presenta oggi in quest'Aula è particolarmente congeniale, che tra i nodi essenziali che il Governo Berlusconi si è impegnato ad affrontare e risolvere con priorità, oltre a quelli della sicurezza e dell'alleggerimento del carico fiscale, campeggia l'infrastrutturazione del Paese. L'Italia soffre, infatti, tutt'oggi di una situazione di arretratezza infrastrutturale che penalizza anche quelle Regioni che maggiormente contribuiscono allo sviluppo economico e che necessiterebbero, invece, di una rete infrastrutturale in grado di garantire, al pari dei concorrenti partner europei, una rete di collegamenti stradali e ferroviari moderna e capillare. di vista posso garantire che lo sforzo per il completamento delle opere necessarie sarà al primo posto dell'agenda non solo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche di tutto il Governo per assicurare quella sinergia indispensabile per il raggiungimento di tale scopo. Alcune delle questioni sollevate nelle interrogazioni sono oggi all'attenzione delle istituzioni europee, mentre altre sono in fase di esame da parte del Parlamento. In entrambi i casi il Governo opererà con impegno per rappresentare gli interessi nazionali e per portare a termine il lavoro sin qui svolto. Fatta questa premessa, che spero possa tranquillizzare i senatori interroganti circa circa le intenzioni del Governo, passo ad illustrare la situazione, ad oggi, delle diverse opere oggetto delle quattro interrogazioni: il nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno, il passante autostradale nord di Bologna, il sistema ferroviario metropolitano e la metrotranvia di Bologna. Chi non è passato per queste strade? il nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno, di cui all'interrogazione 3-00009, preso atto della necessità di risolvere il grave problema infrastrutturale e di viabilità localizzato nella direttrice di attraversamento della città di Bologna,

tra gli «ulteriori interventi di legge obiettivo», nonché nel DPEF 2008-2011. Il nodo riguarda la realizzazione di un'ulteriore variante all'attuale tracciato della strada statale con un itinerario esterno alla perimetrazione del centro abitato del Comune di Casalecchio, che si sviluppa per circa quattro chilometri. Il relativo progetto preliminare, come noto agli interroganti, è stato approvato con delibera CIPE n. 81 del 29 marzo 2006, per un costo delle opere di 147,36 milioni di euro, dei quali 48,86 a carico della rete ferroviaria italiana. Tra gli interventi previsti in legge obiettivo non era stato tuttavia incluso il nodo di Rastignano, cui gli interroganti fanno riferimento. Nelle more della realizzazione del tratto di strada statale 64 Porrettana nel Comune di Casalecchio si è altresì convenuto di realizzare un casello autostradale provvisorio di sola entrata in direzione nord, al fine di ridurre il percorso del traffico locale verso Bologna e, al contempo, di utilizzare quanto più possibile il tratto della nuova Porrettana già realizzato nell'ambito dei lavori della variante di valico. Pertanto, in seguito a precise disposizioni impartite dall'ANAS, la società concessionaria ha assunto l'impegno di costruire il nuovo accesso autostradale. Il relativo progetto è attualmente in fase di istruttoria da parte degli enti che devono rilasciare il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di servizi. Le opere stradali costituenti il nodo ferrostradale di Casalecchio, inclusi gli interventi relativi alla Nuova Bazzanese, sono state inserite nello schema di convenzione unica, redatto ai sensi dell'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni. II suddetto schema è stato firmato in data 12 ottobre ultimo scorso dall'ANAS Spa e dalla società Autostrade per l'Italia Spa In tale schema di convenzione unica è stato inserito l'obbligo, per la società concessionaria, di sviluppare la progettazione del potenziamento di alcune tratte autostradali, tra le quali il nodo stradale di Casalecchio. Tuttavia, come è noto, l'*iter* procedurale di perfezionamento della suddetta convenzione unica non è stato completato nella trascorsa legislatura. Per questo motivo, stante l'urgenza di procedere con rapidità all'approvazione dell'atto convenzionale e al fine di corrispondere alle pressanti richieste di chiarimento da parte delle istituzioni europee in merito al regime delle concessioni autostradali, il Governo ha presentato un apposito emendamento alla legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, che dispone l'approvazione degli schemi di convenzioni già siglati con le diverse società concessionarie autostradali tra cui, appunto, quello con Autostrade per l'Italia. Con l'approvazione definitiva da parte del Parlamento di tale decreto si potrà dare avvio a tutte le opere previste nel suddetto atto convenzionale, tra cui - appunto - il nodo di Casalecchio di Reno.

indirizzata alla Commissione europea-Direzione generale mercato interno e servizi, il Ministro delle infrastrutture *pro tempore* ha formalmente chiesto il parere preventivo sulla possibilità di realizzare lo spostamento di un tratto dell'infrastruttura autostradale (A14) gestita dalla società Autostrade per l'Italia (ASPI) più a nord dell'attuale tracciato, declassando al contempo quest'ultimo a sistema viario locale di scorrimento, con affidamento della relativa costruzione e gestione direttamente all'ASPI. In sostanza, il parere si fonda sulla considerazione che trattasi di variante del tracciato e non di una nuova opera autostradale, il cui affidamento in concessione richiederebbe una procedura di gara, come previsto dalle norme nazionali e comunitarie. Tale richiesta è tuttora all'attenzione della Commissione europea, né sono emersi ulteriori elementi a riguardo nell'ultimo incontro tenutosi il 19 marzo scorso presso i competenti servizi comunitari. Fermo restando l'esito del parere richiesto alla Commissione europea, si ritiene opportuno procedere nella direzione sin qui intrapresa, considerato anche che l'opera ricade tra le infrastrutture prioritarie individuate nell'Allegato 1 al DPEF relativo agli anni 2008-2011 e che, al riguardo, sono state già stanziate dalla legge finanziaria 2008 le risorse necessarie per la copertura degli oneri di progettazione del passante in questione.

di cui parimenti i senatori interroganti chiedono, si deve comunicare che non è stato dato seguito alle iniziative a suo tempo intraprese ai fini della direttiva 2006/38/CE (la cosiddetta direttiva Eurovignette), in quanto la stessa risulta attualmente essere in corso di modifica presso i competenti organismi comunitari. Si è pertanto attualmente in attesa di conoscere le modifiche che verranno apportate previste per il prossimo mese di giugno. Circa Circa l'accordo sul sistema ferroviario metropolitano di Bologna siglato il 19 giugno del 2007 da parte dei rappresentanti del Gruppo FS, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Bologna, come aggiornamento dei precedenti accordi sul servizio siglati nel 1997, Ferrovie dello Stato Spa ha fornito un prospetto riepilogativo che riporta i vari scenari di quel che riguarda gli impegni economici da finanziare, che si rimette a disposizione dell'Aula per la consultazione.

quanto riportato nell'interrogazione in argomento in merito alle fasi approvative e di assegnazione dei contributi, si fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato coinvolto in una prima fase sull'istruttoria del progetto preliminare finalizzata all'assegnazione dei finanziamenti. In tale contesto sono state formulate alcune prescrizioni recepite nella delibera CIPE del 29 luglio 2005 da ottemperare nella elaborazione delle successive fasi progettuali. Attualmente, il progetto definitivo della prima tratta della metrotramvia è stato trasmesso in data 28 gennaio 2008 dal Comune di Bologna, quale soggetto aggiudicatore, al Ministero delle infrastrutture, struttura tecnica di missione per le procedure previste dalla legge obiettivo. Il completamento della documentazione è stato, quindi, effettuato in data 23 aprile ultimo scorso e, pertanto, si prevede di convocare la Conferenza dei servizi già nella

per queste zone; in realtà, si potrebbe chiedere chi di noi non sia rimasto bloccato in questi snodi di traffico. In realtà tutta Italia rimane bloccata

In questi periodi, il nodo di Bologna diventa un groviglio totalmente inadeguato per un Paese avanzato come il nostro. Do atto al Governo della prontezza con cui ha risposto alle nostre sollecitazioni. Intendo la risposta del Sottosegretario come un impegno a tenere monitorati costantemente in sede di Unione europea quei provvedimenti che hanno bisogno di un parere comunitario. Le

sono stati intesi più come interventi di scala locale che non per l'importanza strategica nazionale che rivestono. corridoio tra Berlino e Palermo (il Corridoio europeo 1) eliminando questo intoppo clamoroso nel nodo di Bologna vuol dire fare cose importanti per la modernizzazione del Paese; queste sono infrastrutture relativamente poco costose, ma capaci di dare con molta rapidità forza ad una traiettoria di sviluppo, di modernizzazione e di cambiamento. Prendo atto dell'attenzione e debbo dire che rimango con una preoccupazione che penso di poter esprimere proprio a nome delle nostre comunità: temo che una volta individuati nei diversi settori i punti si trovino poi con altrettanta determinazione non soltanto le risorse ma anche le modalità ed i soggetti per l'attuazione di

locali come una di quelle infrastrutture che potevano essere sostenute attraverso l'intervento del *project financing*, quindi con una modalità che gravasse poco sulle casse pubbliche e che fosse più capace di organizzare investitori e soggetti al fine di una più rapida

banalizzate, quindi con traffico normale. È indispensabile che vada avanti il sistema ferroviario metropolitano, abbiamo già avuto modo per altro di discutere anche in questi giorni (per me è un esordio al Senato) di quanto sia importante

in questo caso completare davvero l'*iter*, perché siamo di fronte ad un processo di realizzazione di queste infrastrutture, che vanno però completate, perché non vorrei che rimanessimo in una condizione per così dire italiana, per cui si fanno le cose a metà o a tre quarti, che poi è come non averle fatte. Per il resto, c'è un intervento in sede comunitaria che auspicabilmente possiamo sostenere e potremmo dare al Governo anche da parte della nostra comunità locale tutto l'appoggio ed il supporto per sostenere in quella sede gli interventi necessari a sbloccare